deputati. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Abbiamo tentato, con l'istituzione della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, di dare una risposta a questo dramma che vive il Paese.

Signor Presidente, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, e soprattutto in Aula, si sono confrontate due linee.

molti emendamenti soppressivi), la quale, al fine di rientrare nei parametri di Maastricht e per affrontare la manovra di politica economica per il 2007, propone un intervento sulla spesa. La proposta è, cioè, che questo rientro avvenga con un taglio lineare degli stanziamenti di spesa corrente,

in una serie di indicazioni specifiche che prevedono diversi tagli che riguardano, com'è tradizione nella proposta politica della Casa delle Libertà, un intervento sulle cooperative, la riduzione di contributi in favore degli enti e delle istituzioni una serie di tagli sulla cooperazione, sul Fondo unico per lo spettacolo, sui servizi di trasporto pubblico e sui servizi di controllo all'interno dell'amministrazione. In aggiunta, si prevede anche di sopprimere autorizzazioni di spesa previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, per il finanziamento dei nuclei di valutazione e verifica sugli investimenti pubblici, sul coordinamento e sull'attività del CIPE. La linea prevede anche una serie di interventi (che non richiamo è uno, particolarmente importante, che dispone il taglio del 90 per cento degli stanziamenti iscritti a bilancio per il trasferimento alle imprese.

ai problemi che sono dinanzi a noi e che sono legati allo sviluppo del Paese, al finanziamento delle opere infrastrutturali e alla realizzazione di misure a sostegno della competitività e delle imprese, coordinandole anche con dei primi passi importanti sul terreno dell'equità. Si tratta di una proposta di carattere alternativo che ha una sua logica, ma che a nostro modo di vedere è sbagliata, perché affida al mercato le possibilità

emendamenti che sono chiaramente soppressivi, mentre abbiamo colto e abbiamo guardato con attenzione ad alcuni emendamenti che contengono delle proposte emendative e che sono indirizzati a realizzare o ad aggiustare

che riguardano l'azione di contrasto all'evasione fiscale e alle iniziative specifiche sulla riduzione dell'area di elusione fiscale; si riferiscono, in particolare, al problema di un rapporto costruttivo con gli intermediari fiscali per ridurre l'area dell'evasione fiscale. Non ignoriamo che su tali proposte vi siano anche delle sollecitazioni che meritano attenzione. sottolineato di tener conto dei tempi ristretti con i quali si affronta la discussione e abbiamo proposto che alle questioni più importanti sia data una prima risposta con la presentazione e l'approvazione di ordini del giorno impegnativi, limitati ad alcune questione essenziali.

accogliere quegli ordini del giorno e di non approvare né gli emendamenti soppressivi, né gli altri emendamenti che hanno caratteristiche più circoscritte.

che hanno aspetti di carattere strutturale, rappresentati dal rafforzamento della riforma della riscossione. ricordare che oggi per i contributi previdenziali e per i tributi fiscali opera una società, la Riscossione costituita nell'ultima fase del Governo precedente, con la legge finanziaria del 2006. In continuità con quella riforma, noi i poteri, perché il problema della riscossione è decisivo per implementare le risorse e per realizzare un'operazione graduale di rafforzamento delle entrate.

che oggi tutti conosciamo, in base alle quali i quartieri centrali pagano meno ICI rispetto a quartieri

per contrastare e ridurre al minimo le frodi nel campo dell'IVA e per permettere, in tempo reale, all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza

delle entrate fiscali è il risultato di un incremento del PIL

In continuità con quelle misure, tendiamo a rafforzare di molto l'attività di monitoraggio, che rappresenta l'attività preventiva. Ricordiamo che le maggiori entrate non sono l'effetto del condono: la politica dei condoni, poi abbandonata nell'ultimo anno e che noi respingiamo, è stata sciagurata. Mi spiego: i condoni sono stati fatti in maniera anonima. E questo fino al 2003 lega le mani all'amministrazione fiscale ed alla Guardia di finanza che non sono in grado di fare una azione intelligente. condoni, inoltre, sono stati strutturati per la parte più consistente con una singolare decisione: quella che l'effetto ai fini penali e fiscali, cioè l'effetto tombale, decorreva già dal pagamento della prima rata. Cosa è avvenuto?

del giorno che abbiamo presentato, alcuni di merito: uno relativo al problema delle successioni e delle donazioni, dove poniamo il problema di estendere la franchigia ad una platea più vasta di cittadini perché ci sembra troppo limitata l'attribuzione di quella franchigia solamente al coniuge, ai figli, ai nipoti. Chiediamo poi di chiarire fino in fondo che non devono esserci effetti nel passaggio generazionale di azienda,

approvate alla Camera sulla deducibilità dell'auto e chiediamo anche un'attenzione alle modifiche antielusive sui problemi del catasto. A ciò si aggiungono altri due ordini del giorno che riteniamo di grande valore. Il primo, veniva ricordato ieri in conclusione del dibattito anche dal presidente Morando,

devono essere utilizzati per ridurre le tasse, a partire dai redditi più bassi, delle famiglie e delle imprese. Si tratta, quindi, di finalizzare la lotta all'evasione fiscale. In conclusione,

Lo Statuto è stato definito con un lavoro comune di tutto il Parlamento ed è alla base di un rapporto moderno nella società di oggi,

i commercialisti, i ragionieri, i tributaristi, i diversi ordini professionali ed i CAF. Sappiamo che la concertazione non può significare contrattazione, ma sappiamo anche che essa deve significare considerazione delle ragioni, delle proposte e delle necessità, anche di gradualità, con le quali le nuove tecnologie debbono essere adottate.

e generale; non ci sono - lo avvertiamo fortemente - ragioni di equità, ma chiudere gli occhi, rinviare alle calende greche e fare proposte che non stanno in piedi sull'evasione fiscale significa commettere anche altri errori. Primo errore: come possiamo parlare di economia e di mercato in presenza di evasione fiscale, un forte fattore di perturbazione della concorrenza? Come possiamo dare una risposta ai problemi della professionalità, dell'impegno sul lavoro, della capacità di rischiare per intraprendere se poi abbiamo il lavoro sommerso e l'evasione fiscale? Come possiamo ridurre le tasse in maniera significativa se l'evasione fiscale non viene contrastata? Forse ponendo in essere altre soluzioni che sembravano semplici ma non hanno funzionato come quella di ridurre le tasse

efficiente ed efficace alla ripresa del nostro Paese e ad una operazione in cui la crescita si coniuga con il rigore e con l'equità.

e, purtroppo, non si è riusciti a svilupparlo ulteriormente in Aula. La tesi che era stata ampiamente articolata in Commissione e che è riecheggiata nei pochi interventi in Aula, relativamente all'impostazione e all'ispirazione di questo provvedimento, è la seguente: voi avete impostato una manovra fondata sull'aumento delle imposte e della pressione fiscale, mentre noi avremmo provveduto a ridurre le spese. Tale tesi viene sostanziata anche attraverso le coperture recate dagli emendamenti presentati dalle opposizioni.

e lo abbiamo fatto sostenendo - richiamo soltanto per titoli gli argomenti - che è vero che la pressione fiscale aumenta ma in modo contenuto per il prossimo anno, e inoltre aumenta in misura inferiore a quanto sta avvenendo nel corso del 2006 per effetto

riduzione della pressione fiscale. L'aumento leggero, contenuto ma necessario della pressione fiscale, dunque, è da considerarsi transitorio e temporaneo. Abbiamo detto e ribadiamo che le riduzioni di spesa nell'impianto complessivo della manovra ci sono, sono realistiche e rappresentano una parte corposa della manovra stessa, cioè circa 11 miliardi di euro, appostati nei principali capitoli di bilancio. Le opposizioni non hanno risposto a queste tesi nel merito ma hanno solo ribadito la loro posizione asserendo che le riduzioni indiscriminate di spesa sarebbero la via per via per completare il percorso di risanamento. Sennonché la loro tesi è contraddetta dai risultati che in questi anni sono venuti dalle politiche economiche e di bilancio. Soprattutto nell'ultimo anno, il passato Governo ha realizzato tagli indiscriminati che sono risultati totalmente inefficaci e non hanno dato

del dissanguamento delle casse dell'ANAS (che ha determinato il blocco dei cantieri), della decozione delle ferrovie (alla quale stiamo assistendo in queste settimane e alla quale bisognerà porre rimedio), delle difficoltà di molti settori importanti della pubblica amministrazione (la sicurezza, la giustizia, la scuola ed altro). Abbiamo voluto dare un approccio serio, realistico; abbiamo individuato, con il DPEF, le quattro macroaree di spesa sulle quali intervenire. Su due di queste stiamo stiamo intervenendo già con questa manovra: mi riferisco alla sanità, attraverso la stabilizzazione della spesa e il taglio della spesa tendenziale, e agli enti locali, attraverso la redazione del nuovo patto di stabilità. Lo faremo Lo faremo per il sistema pensionistico, con la riforma concertata che dovrà avviarsi a partire dal mese di gennaio, e per il pubblico impiego, con la riforma della pubblica amministrazione, anch'essa in fase avanzata di elaborazione. elaborazione. Bisognerà intervenire ancora. I risparmi possono venire anche da molti altri settori: dal completamento delle liberalizzazioni, dalla riforma dei servizi pubblici locali ed altro. È certo che continuare a tagliare con l'accetta, in modo indiscriminato, non risolve i problemi, introduce iniquità, produce disservizi ed inefficienze - che ho richiamato - e molto altro. Il senatore Menardi ha detto testualmente che il Governo non capisce che il vero problema è la crescita. Certo che lo capisce, collega Menardi. Non solo l'obiettivo della crescita economica è uno dei tre obiettivi fondanti dell'intera politica economica, così come disegnata nel DPEF, ma, anzi, essa ne costituisce l'asse centrale, con le proposizioni che sono state avanzate in quel documento, con questa manovra e nella discussione che abbiamo tenuto. In base a tali proposizioni, senza il risanamento non è possibile una crescita stabile e duratura; e l'equità sociale, che vogliamo introdurre e che già introduciamo con questa manovra, non soltanto è giusta ed è un valore in sé, ma aumenta la domanda (quantomeno per beni di consumo) e quindi sostiene, per questa via, la crescita economica. Sulle misure di contrasto all'evasione e all'elusione ha già parlato il presidente

si introducono troppi poteri straordinari, che vi è un approccio invasivo (il Grande fratello richiamato dal senatore Ciccanti in questa discussione) ed altri argomenti che abbiamo ascoltato. È vero - come ha detto il collega Ripamonti - che la discussione sulla*privacy*, sulla valutazione di questi strumenti introdotti, è seria. È vero che l'aumento della pressione fiscale - come ho già accennato - non è utile alla crescita; lo ha spiegato in modo efficace il presidente Morando. È vero che lo statuto del contribuente va rispettato; lo abbiamo detto nella discussione, ha detto il presidente Benvenuto e lo abbiamo affermato in un ordine del giorno. Ma noi abbiamo assunto due impegni forti su questo terreno. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: l'aumento della pressione fiscale è temporaneo vorremmo destinarne i maggiori proventi alla riduzione della pressione fiscale, già a partire da una norma da introdurre nell'articolo 1 della finanziaria. costituisce l'oggetto di un ordine del giorno approvato in Commissione, che vorremmo tradurre, appunto, in norma giuridica da inserire nella legge finanziaria, a partire da quest'anno. In ogni caso, le misure che costituiscono l'oggetto del decreto-legge sono normali e civili. Pensate al tema delle compensazioni: come si può sostenere che se un settore della pubblica amministrazione è creditore nei confronti del contribuente e chiede quindi di poter compensare il debito erariale con il credito, ciò costituirebbe una vessazione? Non è affatto vero.

Vi prego. Vada avanti, senatore. inaccettabili e straordinari, quando le garanzie processuali rimangono assolutamente intatte? Sono argomenti per lo più pretestuosi, a volte totalmente distanti dal contenuto effettivo delle norme che sono state emanate. Sulla seconda parte del decreto - mi avvio a concludere - è stato detto poco in questo dibattito. Vi è stato un solo riferimento - quello del senatore Saro - alla riforma del rapporto ANAS - società concessionarie (i commi 82-90), norme ampiamente spiegate e commentate, quanto alle ragioni ispiratrici e ai contenuti, dalla presidente Donati. Sul punto volevo ulteriormente intervenire per fare alcune precisazioni utili - mi auguro - al prosieguo del confronto. Che i rapporti in essere tra ANAS e società concessionarie non funzionassero è pacifico

Pertanto, che occorresse intervenire normativamente non può essere opinato. Certo, era ed è difficile contemperare l'interesse pubblico, quello all'effettiva realizzazione degli investimenti e al contenimento delle tariffe, con interessi e diritti consolidati, nei contratti che accedono alle concessioni. Era ed è un compito molto difficile.

che permangono. È di questa mattina la notizia che il tribunale di Genova ha rimesso alla Corte di giustizia la questione relativa alla compatibilità tra la suddetta normativa e i principi comunitari. Noi ci siamo anche impegnati con un atto ben preciso, un ordine del giorno discusso approfonditamente, ad apportare nel futuro (anche nell'immediato futuro) gli adeguamenti necessari, sulla base delle indicazioni dell'Unione europea, a introdurre un soggetto terzo che possa coadiuvare la regolazione dei

anche nel prosieguo della discussione con l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Intanto, il decreto va approvato, le risorse finanziarie che esso reca devono essere certe, perché è necessaria la manovra nel suo complesso. Le misure introdotte sono importanti e vanno approvate. Occorre che conseguiamo rapidamente maggiori certezze maggiori certezze nello svolgimento della sessione di bilancio, attraverso la rapida, definitiva e completa approvazione di questo decreto. Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di entrare nel merito del mio intervento, desidero ringraziare a nome del Governo i due relatori, il senatore Legnini e il senatore Benvenuto, i quali hanno illustrato, prima in Commissione e poi in Aula, il provvedimento che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea del Senato. Un ringraziamento va esteso a tutti i senatori che sono intervenuti prima in Commissione e poi in Aula per gli importanti contributi che sono stati apportati al dibattito, dei quali il Governo terrà debitamente conto nel corso della discussione sulla legge finanziaria che si svolgerà nelle prossime settimane in Senato. Nel corso del dibattito è stato posto l'accento sul carattere di collegamento non solo formale, ma anche sostanziale che ha il provvedimento in esame, finalizzato alla copertura della manovra finanziaria per il 2007, con il quale si anticipa di fatto la discussione sulla sessione di bilancio. Questo dato ha indotto legittimamente i senatori intervenuti a svolgere, insieme all'esame puntuale dei contenuti del decreto, considerazioni sul complesso della manovra approvata dalla Camera, sugli effetti che essa genera per le prospettive del nostro Paese, anche in relazione agli impegni di carattere europeo che la caratterizzano. Il decreto che è alla nostra attenzione ha un collegamento naturale con il decreto sulla liberalizzazione e sulla concorrenza approvato lo scorso luglio ed è coerente con gli obiettivi principali riassunti dalla manovra: obiettivi di risanamento, crescita ed equità. Vorrei partire da un punto centrale del decreto, che è stato sottolineato poc'anzi anche nelle conclusioni del senatore senatore Benvenuto. È un tema sul quale è importante che si concentri l'attenzione del Parlamento e del Paese, vale a dire la lotta all'evasione fiscale. La proposta contiene un'articolazione di misure particolarmente importanti a sostegno dell'attività di prevenzione e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, che, com'è noto a tutti, hanno raggiunto un'entità quantificata dall'Agenzia delle entrate un importo assolutamente intollerabile per un Paese moderno e civile. Si è deciso, quindi, di intervenire su questo punto in maniera efficace e strutturata, rafforzando gli strumenti e le procedure dell'accertamento, anche attraverso un utilizzo più incisivo degli strumenti e delle tecnologie informatiche, agendo sul rafforzamento dell'azione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, rafforzando il ruolo e la funzione dell'Agenzia delle dogane prevedendo ulteriori misure in materia di riscossione, il cui ritorno in mano pubblica, operato dal precedente Governo, entra a regime in maniera definitiva. Questo complesso di misure sarà accompagnato da un'attenzione specifica al tema del miglioramento del rapporto tra amministrazione fiscale e cittadini, argomento sul quale il Governo è consapevole di dover investire un'attenzione e una volontà superiori a quelle manifestate fin ora. In questo senso va anche la costituzione della Consulta, alla quale faceva riferimento poc'anzi in conclusione il relatore. al tema dell'evasione molti senatori hanno giustamente dedicato la loro attenzione e avanzato una sollecitazione, contenuta in uno degli ordini del giorno accolti dal Governo nei lavori delle Commissioni 5ª e 6ª, cioè quello di utilizzare le risorse provenienti dal recupero dell'evasione per ridurre la pressione fiscale su famiglie ed imprese. «In ragione di ciò, il Governo sarà impegnato a presentare, a decorrere dal 30 giugno 2008 e successivi, un documento di rendiconto sugli effetti dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, e a valutare l'opportunità di destinare le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a quelle preventivate dal bilancio, destinate a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità e crescita che lega il Paese agli altri Paesi dell'area euro e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economica e finanziaria, alla riduzione della pressione fiscale raggiunta nel 2007». Ho citato integralmente il dispositivo di uno dei diversi ordini del giorno che sono stati accolti per testimoniare il valore che abbiamo voluto attribuire alla discussione avvenuta in Commissione, nella quale abbiamo manifestato in modo assolutamente trasparente la volontà di approvare il decreto fiscale senza modifiche, ma di tradurre in emendamenti alla finanziaria gli argomenti accolti in sede di Commissione dal Governo. I relatori prima e poi, nel corso del dibattito, altri interventi hanno posto in evidenza gli altri aspetti salienti del decreto su diverse materie, le cito per titoli e non tutte: il catasto, per il quale è prevista una delega al riordino (vengono trasferiti in questo modo i comuni strumenti di riordino e d'equità), si è poi precisata la disciplina d'intervento per quanto riguarda gli immobili in classe A ed E, altre misure riguardanti l'IVA, la tassa sulle successioni, gli interventi in materia di infrastrutturazione e in relazione alle decisioni riguardanti lo Stretto di Messina, ANAS e Autostrade, l'editoria ed un complesso di altri La discussione che si è svolta sinora ha fatto emergere delle criticità su aspetti non sempre marginali dei singoli argomenti trattati. Il Governo ha seguito - credo di poterlo dire - con serietà e attenzione questo dibattito e in conclusione ritiene di dover confermare, insieme alle determinazioni già comunicate in sede di votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, alle Commissioni riunite 5a e 6a , la disponibilità ad approfondire i temi che non hanno trovato una compiuta definizione in questo decreto. Mi riferisco al tema delle donazioni e delle successioni, all'IVA detratta sulle auto aziendali, all'esigenza di approfondire la norma concernente le concessioni autostradali, alla coerenza dei provvedimenti con il dettato dello Statuto del contribuente, alle norme riguardanti l'editoria e ad un complesso di altre questioni.

dell'entità della manovra che proponiamo all'attenzione del Parlamento e concludo il mio intervento invitando il Senato a dare il consenso al provvedimento che viene sottoposto all'esame e all'approvazione nella seduta odierna.

affatto convinto sui buoni fondamenti di questo decreto, sulla sua legalità, sulla sua necessità, sulla sua giustezza e quindi sul perseguimento di quella proporzionalità che sappiamo deve essere misurata tra le disposizioni introdotte e i diritti del cittadino.

il provvedimento reca delle norme contrarie alla legge di contabilità; ricordiamo - lo sanno benissimo i colleghi, perché tante volte ne abbiamo parlato - che la legge di contabilità è un provvedimento che, rispetto alla legge ordinaria, gode di una resistenza passiva superiore, e quindi non è paragonabile alle altre leggi coordinate, in quanto sappiamo che la legge di contabilità può essere modificata soltanto da leggi che non siano la legge finanziaria e la legge di bilancio né i provvedimenti collegati. Per l'appunto, nella legge di contabilità è previsto che i provvedimenti collegati dispongono dell'acquisizione delle rinvenienze di risorse che non possono essere utilizzate nella finanziaria e, al loro interno, devono avere natura di omogeneità.

ma proprio in funzione del suo collegamento dovrebbe avere natura omogenea e le risorse rinvenienti dal provvedimento non potrebbero essere utilizzate come fonte di copertura della finanziaria. finanziaria. La Commissione bilancio ha aggirato la dichiarazione di collegamento che codesta Presidenza ha fatto, dicendo che il provvedimento non è un collegato *ex lege* di contabilità, ma è un collegato di tipo politico. Ma perché questo non può soddisfarci? perché il collegamento politico non era stato chiesto, anzi tutt'altro, era stato negato dalla risoluzione che approvava la Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria e che il precedente citato, e cioè il fatto che alla Camera il collegamento sia stato non giudicato dalla Commissione bilancio, non può fare precedente per questo ramo del Parlamento, perché al contrario, nel passato, le dichiarazioni non avevano costituito precedente per la non dichiarazione di collegamento in questo ramo del Parlamento. Ma perché è importante ancorché dal punto di vista formale, da quello sostanziale, la dichiarazione di collegamento? Perché così, la contrarietà alla legge di contabilità risulta evidente in quanto la manovra finanziaria non è considerata dai due rami del Parlamento in modo unitario per affrontare quei problemi riguardanti

che espungono la realtà e la sostanzialità della legge finanziaria di modo che quest'ultima verrebbe ad essere prodotta soltanto per articolo 1, vale a dire per l'ammontare dell'indebitamento, cioè per il fabbisogno e quindi per l'emissione di BOT.

al Paese, intaccando il risparmio del cittadino. Ebbene, noi sosteniamo che la proprietà non è un furto e che il risparmio è una riserva non aggredibile, che

una delle fonti di copertura essenziali della legge finanziaria. A sua volta, in questo provvedimento le norme di maggior rilievo sotto il profilo delle entrate sono quelle relative alla lotta all'evasione fiscale.

per la maggior parte permanenti e dunque crescenti. Non ci nascondiamo che gli effetti di cassa previsti nel decreto-legge sono di gran lunga inferiori a quelli di competenza, perlomeno nel primo periodo. Tuttavia,

signor Presidente, potrebbe dare origine ad una scopertura sostanziale del decreto-legge e dunque della legge finanziaria. Come si comprende, gli effetti potrebbero essere davvero gravi

favorire l'emersione del sommerso attraverso una riduzione della pressione fiscale, si è rivelata vincente. Ancora oggi in Commissione bilancio stiamo esaminando una cifra che a lungo non è stata citata nel dibattito sulla finanziaria: il risparmio pubblico di oltre 22 miliardi di euro che questo Governo si Tutta la drammatizzazione iniziale era priva di fondamento. C'è stato un miglioramento del risparmio pubblico di 22 miliardi di euro provenienti da maggiori entrate, frutto di una politica, antitetica a quella posta in essere finanziaria, che riduceva le aliquote per aumentare la base imponibile dando vita ad un circolo virtuoso delle imposte: minor peso su ciascuno, maggiore estensione della base imponibile.

probabile di una scopertura evidente di questa legge finanziaria, che attraverso un circolo vizioso finanzia le uscite, maggiori spese permanenti, strutturali e crescenti, con maggiori entrate eventuali ed incerte. Nei consuntivi potremo trovarci, come già è accaduto per altre imposte, di fronte a veri e propri buchi di bilancio, tenendo presente che questo pericolo può diventare addirittura

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene di richiedere il non passaggio agli articoli. Facciamo questo, presidente Marini, perché non possiamo

assurdo ed evidentemente la Giunta per il Regolamento dovrà, a mio avviso, pronunciarsi perché, per una serie di motivi che seppure sinteticamente voglio elencare, mi pare veramente assurdo non poterlo fare.

l'attuale Presidente della Repubblica ha ritenuto di comportarsi in maniera diversa e non vogliamo certamente aprire una polemica con il Capo dello Stato, però questo è un dato di fatto.

novembre, cioè pochi giorni fa, il tribunale di Genova ha deciso di presentare ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 del Trattato dell'Unione Europea. Il ricorso trae origini dal contratto-convenzione stipulato il 27 settembre tra Consel-GMFR e la Slala; praticamente si tratta della realizzazione del Terzo valico. Ora, il decreto non è ancora convertito in legge e già un tribunale chiede di consentire

di individuare - non soltanto il Gruppo UDC, ma credo anche altri colleghi dell'attuale maggioranza - circa l'attuale Regolamento del Senato e l'attuale legislazione, che riguarda

Il collega Matteoli molto opportunamente ha fatto presente che siamo in qualche misura indotti o persino costretti a votare il non passaggio all'esame degli articoli, che è una votazione che di per sé fa cadere l'intero provvedimento, perché non vi è la possibilità dello stralcio, trattandosi di decreto-legge.

Chiedo scusa perché è una questione di carattere procedurale e che richiede anche un'attenzione degli Uffici.

un'utilizzazione di strumenti parlamentari diversi rispetto al non passaggio all'esame degli articoli, pensando, per esempio, che si possano colpire singole parti dei provvedimenti di urgenza, dei decreti-legge? È questo un consiglio che do alla Presidenza del Senato, ma che finisce per essere un consiglio al Governo

siamo consapevoli che si tratta di una procedura estrema rispetto all'intendimento reale, che è quello del confronto parlamentare sul merito. Allora, se la regola è il confronto parlamentare, se non vi è il voto di fiducia su singoli provvedimenti e se non vi è un uso improprio dello strumento della decretazione di urgenza da parte del Governo, ovviamente il confronto parlamentare diventa la regola istituzionale nuova come tale, prevalente rispetto agli strumenti parlamentari che si può essere costretti ad utilizzare di fronte all'inesistenza di questa regola. Capisco che diventa forse impossibile chiedere al Governo un impegno a non porre mai la questione di fiducia in via di principio (vi possono infatti essere circostanze che lo richiedono), ma, di fronte ad un'intesa istituzionale che comporta la possibilità concreta di votare alcune parti dei provvedimenti (e non quindi di non votare per niente), di fronte al non uso ostruzionistico della procedura parlamentare, non è possibile cercare un'intesa istituzionale, della quale il Senato si possa far carico, per esempio, in materia di finanziaria e di decreti-legge, stabilendo che, se essa prevale, le condizioni sono che non vi sia un numero eccessivo di emendamenti, che non si ponga la questione di fiducia e che il decreto‑legge non contenga elementi impropri? Ciò che intendo dire è che l'intesa istituzionale non è soltanto la legge elettorale o la riforma costituzionale, ma è gran parte della vita politica quotidiana. In questo caso, il Gruppo di opposizione dell'UDC ritiene di essere costretto a far ricorso ad uno strumento eccessivo rispetto agli intendimenti perché manca una procedura parlamentare adeguata ad un'intesa istituzionale che abbia nel confronto parlamentare il punto di merito, di merito, anziché lo scontro parlamentare. Dico questo anche perché, come credo sia stato evidente, l'UDC sta cercando disperatamente,

di valutazione del decreto fiscale, non possiamo che riscontrare più di una necessità del riesame o della riconsiderazione dei termini del decreto.

che le previsioni del nostro Regolamento da applicare a questo decreto siano concretamente evidenti.

nel momento in cui - com'è successo già alla Camera e come succederà senz'altro al Senato - verranno modificati i saldi della legge finanziaria per effetto di un decreto fiscale che molto probabilmente avrà un'incidenza

L'1.100 è uno degli emendamenti a cui l'opposizione attribuisce maggiore importanza perché, di fatto, delinea una manovra radicalmente alternativa a quella proposta con il decreto-legge.

costituisce uno degli elementi portanti di questo provvedimento e della manovra. Poiché intendiamo attribuire a tale proposta l'intento di

un nostro principio cardine, quello di lavorare non sulle maggiori tasse prelevando soldi dei cittadini, ma operando seriamente sulla riduzione della spesa corrente.

eccessivamente o discrezionalmente su un comparto o sull'altro, ma, attraverso una riduzione di assai modesta entità, su un elevato numero di capitoli, riesca invece ad ottenere

minori tasse sui cittadini e dando corso a un processo virtuoso di miglioramento del ciclo economico e della competitività del Paese, che costituiscono i due problemi che abbiamo di fronte e che il Governo non riesce in alcun modo affrontare. Vorrei osservare che il Governo, un po' maldestramente, fa un'operazione simile con l'ex articolo 53 della legge finanziaria (che ora credo sia il comma 206 dell'articolo 16; mi scuso per la non precisione del riferimento, ma la norma l'abbiamo presa in esame solo questa mattina), laddove usa un meccanismo molto tortuoso e molto dubbio sotto i profili dell'aderenza alle norme di contabilità, dire un accantonamento trasversale di fondi (con alcune esclusioni) che a discrezione del Governo, potrebbero poi essere ridotti. Oltre alla discrezionalità assurda e talvolta mortificante (penso all'utilizzo eccessivo del fondo per le aree sottoutilizzate, di nuovo interamente attratto nella discrezionalità del Governo),

oggi deve tendere a migliorarlo. Il Governo e la maggioranza hanno tutto il tempo di migliorarlo in quest'Aula e sottoporlo di nuovo alla Camera per la definitiva approvazione. Per queste ragioni, chiediamo l'accoglimento

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, l'emendamento 1.2, con lo stesso spirito che caratterizza un un insieme di emendamenti presentati da tutta la Casa delle Libertà, mira a denunciare che la manovra è sbagliata e a proporre un'inversione

Abbiamo ritenuto di denunciare che la manovra della maggioranza di centro-sinistra è tutta spostata sul lato delle entrate, come oramai i i commentatori economici e finanziari più avvertiti, lo stesso Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Confindustria e le stesse organizzazioni sindacali hanno rilevato. Non si agisce sul lato dell'offerta: è vero che ci sarà una seconda fase, e la verificheremo, ma certamente, rispetto alle indicazioni del DPEF del luglio scorso, questa manovra

come le cosiddette riforme strutturali agiranno sul lato dell'offerta. Sta di fatto, signor Presidente, che, con questo decreto,

e della legge finanziaria dovrebbero incidere sull'accertamento, mentre è riconosciuto da questa maggioranza, ma anche da Tremonti quindi dalla maggioranza

l'emendamento 1.3 ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una fondamentale disposizione che attiene ai diritti del contribuente e allo stesso tempo alla promozione di una reale collaborazione tra il contribuente stesso e l'amministrazione finanziaria. Una disposizione che è mutuata dal *Taxes* *Management* *Act* del Regno Unito, una legge del 1970 che stabilisce come l'amministrazione finanziaria possa acquisire informazioni su un contribuente soltanto in due, e solo due, fattispecie: quella del fallimento del contribuente stesso o quella che si realizza nel caso in cui il contribuente non dia le informazioni che gli sono state richieste. Anche in questo caso, peraltro, questa disposizione prevede che l'amministrazione debba informare tempestivamente, entro dieci giorni, il contribuente delle informazioni che sono state raccolte sul suo conto. Tale disposizione, ove accolta, avrebbe come conseguenza quella di far decadere numerose delle disposizioni previste dal cosiddetto decreto Bersani-Visco e numerose disposizioni che qui sono esplicitamente indicate, contenute cioè nello stesso provvedimento all'esame. Ricorrentemente e anche in questo provvedimento, infatti, si prevedono modalità di acquisizione di informazioni che escludono il contribuente e soprattutto gli impediscono di poter controdedurre, nel caso in cui egli non ravvisi la correttezza di tali informazioni. ricordare, a tale proposito, che la profonda differenza che si rinviene tra la legislazione promossa da questo Governo e quella del precedente Governo, con riferimento al contrasto dell'evasione, riguarda proprio il rispetto dei diritti del contribuente. Vorrei ricordare, in particolare al presidente Benvenuto, che ha parlato di continuità tra le misure anche qui disposte e quelle già varate nel corso della trascorsa legislatura, ad esempio, del trasferimento di informazioni da parte delle aziende di credito all'amministrazione finanziaria,

include una valutazione assolutamente discrezionale, da parte dell'azienda di credito, sulle ragioni di quella transazione. Rispetto a questa valutazione discrezionale, il contribuente non ha nessuna possibilità di controdedurre e di contestare quelle valutazioni, di cui egli non viene assolutamente a conoscenza. Lo stesso vale per le informazioni estrapolate dalle camere di commercio, ove richiesto di fornirle, o, ancora, per le numerose informazioni che dovrebbero essere richieste ai cittadini cittadini (oltre tutto sanzionate ove non seguite da adeguata risposta da parte del cittadino) su contribuenti che rimangono a lui ignoti. È un modo veramente trasversale dell'amministrazione, non trasparente, che sembra non rivolto all'identificazione delle possibili situazioni patologiche di potenziale evasione, ma che sembra piuttosto rivolto ad acquisire indiscriminatamente informazioni sui contribuenti, sulla base di una sorta di presunzione di colpa del contribuente stesso per il solo fatto di esistere. Anche in questo provvedimento si riproducono modalità invasive dell'amministrazione finanziaria; gli stessi collegamenti telematici, che vengono richiesti nella direzione dal contribuente all'amministrazione, sono in realtà funzionali al percorso inverso, che l'amministrazione ovviamente impiegherebbe per un'intrusione nell'attività quotidiana del contribuente. Ora, noi pensiamo che sia assolutamente fondamentale ripristinare i diritti del contribuente e favorire la leale collaborazione di esso con l'amministrazione finanziaria, quale si è rivelata nei dati che il dipartimento delle entrate ha fornito per quanto riguarda la prima parte dell'anno: quello straordinario più 21 per cento nelle entrate dirette che si è registrato nei primi sei mesi e, ancora, quel più 14 per cento che si è verificato nei primi dieci mesi, che vanno ben oltre l'andamento positivo dell'economia, la pur modesta crescita che si è registrata nel corso dell'anno. Ad indicare che si era innescato un processo virtuoso nel rapporto tra contribuente ed amministrazione, che viene violentemente interrotto dalla costruzione di un odioso Grande fratello fiscale *(Applausi macchina da Stato di polizia tributaria, che può essere fermata, se il Parlamento vuole, semplicemente affermando il fondamentale diritto del contribuente di conoscere le informazioni raccolte dalla macchina pubblica e che lo riguardano; per poter controdedurre in un rapporto trasparente, l'unico che può costituire il concorso di tutti, in un contesto di assoluta equità, alla fiscalità generale.

per quella leale collaborazione tra fisco e contribuente di cui parlavo poco fa. Essa riguarda l'irretroattività sostanziale di tutte le disposizioni fiscali. Era un principio affermato nello Statuto del contribuente e che poi è stato sistematicamente violato dall'attuale Governo

e che sono, quindi, conseguentemente soppresse. Ricordo il comma 18, lettere *b)* e *c)*, in tema di ammortamento dei fabbricati aziendali; i commi da 33 a 36, nonché ai comma 38, l'ultimo periodo, in materia di catasto, terreni e fabbricati agricoli; il comma 43, relativo alle rendite catastali (categoria E); il comma 72, concernente lo speciale regime di disfavore introdotto per le auto aziendali. Sono tutte misure che costituiscono arbitrari interventi retroattivi e che odiosamente cambiano le condizioni

un regime fiscale che viene invece così modificato in corso d'opera. Per non parlare di quella odiosa disposizione che nella versione originaria voleva una pesante sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale in una sola occasione e che poi, opportunamente, è stata corretta chiedendo quale presupposto tre violazioni. tuttavia, ancora incomprensibilmente previsto che il nuovo regime si applichi solo alle violazioni contestate solo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione che stiamo discutendo, mentre il regime previgente, quello dell'unica violazione, continua ad applicarsi per quelle contestate in precedenza. Segnalo ad ogni modo che, quando parliamo di irretroattività sostanziale, ci rivolgiamo a tutti i profili che delineano i tratti essenziali del rapporto tributario, il che significa che ci riferiamo anche all'esercizio della potestà di accertamento svolta dall'amministrazione, che non può in alcun modo ritenersi mera attività procedimentale, insensibile alle garanzie fondamentali del contribuente. Quindi, anche in questo caso, va riaffermato il divieto di retroattività, sanzionato con l'immediata e automatica cessazione di efficacia di tutte le disposizioni contrarie, così da consentire un immediato e non comprimibile effetto percepito da parte di tutti i contribuenti. Signor Presidente, il Santo Padre ci ha recentemente richiamati ai fondamentali della civiltà occidentale, quei fondamentali in nome dei quali non saremmo mai disposti a credere in un Dio irrazionale e discrezionale. Tanto meno saremmo mai disposti a credere in uno Stato che si presenti irrazionale e discrezionale.

Siamo convocati oggi in seduta pubblica e all'ordine del giorno vi è il seguito della discussione del disegno di legge grazie anche all'atteggiamento - spero almeno questo lo riconosciate - positivo della minoranza (ad esempio, il Gruppo di Alleanza Nazionale su 30 emendamenti ne ritira 11) perché vogliamo confrontarci sul merito e non vogliamo darvi alibi per la fiducia.

che recita «Ciascun senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in esso contenute siano stralciati» siano stralciati» non riguarda i decreti-legge. Eppure, stiamo parlando di un disegno di legge che include un decreto-legge.

perché ci sono norme che magari con la ragionevolezza si potrebbero modificare senza che cada il Governo.

ci dovrebbe essere per tutti. STORACE *(AN)*. La seconda questione, che non siamo riusciti a dirimere nel dibattito precedente in merito, era legata ai presupposti di costituzionalità. Il Governo ha stabilito, con la norma che proponiamo di modificare,

necessità e urgenza? Non abbiamo potuto parlarne. La terza questione riguarda l'esame delle pregiudiziali di costituzionalità, che in questo caso riguardano le modifiche che dalla Camera sono intervenute al Senato.

con qualche profilo di dubbia costituzionalità, perché si deve accertare la violazione se poi si vuol far sospendere o chiudere l'attività.

e nell'arco di cinque anni sono pizzicato per tre volte nel non emettere scontrini fiscali, sono praticamente un evasore

se si contestano e non si accertano tre violazioni in cinque anni e non tre violazioni in un mese: lì sì che c'è l'abitudine a violare la legge. Ecco perché vi chiediamo di correggere una norma che sarebbe nel solco di quello che voi avete preannunciato col decreto-legge fiscale. al nostro esame sono un manifesto ideologico di questa maggioranza, è evidente. Si vuole colpire, come nel comma 1, un ceto che non ha votato il centro-sinistra, e mi riferisco ad un dato evidente:

Questa è la vendetta, la criminalizzazione di un ceto sociale che non vi ha votato, e dico anche che è una manifestazione particolarmente odiosa,

in materia di sanzione amministrativa accessoria per la mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscali, che sanciva l'applicabilità delle normali garanzie per il contribuente che volesse impugnare gli atti di accertamento. Si vuole, cioè, reintrodurre il concetto che soltanto dopo l'esaurimento delle normali procedure di impugnazione e quindi soltanto in presenza del definitivo

non intacca solamente i princìpi dello statuto del contribuente, princìpi che peraltro dobbiamo riconoscere applicati dai servizi ispettivi della Guardia di finanza e dagli uffici ispettivi delle Entrate, ma non certo da questo Governo. Questo Esecutivo sembra non riconoscere che lo statuto del contribuente è stata approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento e non solamente dalla maggioranza di Governo precedente.

le nostre valutazioni sull'intero articolo 1. articolo 1. Colleghi senatori, poiché il presidente Marini ha giudicato questo provvedimento come formalmente collegato alla finanziaria, abbiamo il dovere di svolgere le nostre riflessioni nel pacchetto complessivo della manovra di politica economica che il Governo ci sta presentando, oggi con il cosiddetto decreto fiscale e la prossima settimana Signor Presidente, onorevoli colleghi, è in atto un'operazione che, se fosse svolta da un normale consiglio di amministrazione di una qualunque società per azioni italiana, vieppiù se quotata in Borsa, configurerebbe il reato di false comunicazioni sociali. In base a quello che ho ascoltato sia in Commissione sia in Aula stamattina, questo ramo del Parlamento sta procedendo a varare un provvedimento che contiene appunto il reato di false comunicazioni sociali; false in termini di realtà economica che viene a prodursi sull'economia italiana a seguito di questo decreto e della legge finanziaria e false in rapporto alle condizioni tra Stato e cittadino che vengono a determinarsi con il decreto in esame e con la finanziaria. In termini di realtà economica, è già stato detto da altri colleghi dell'opposizione, vi è una diversa impostazione tra questa maggioranza e questa opposizione. È stato detto che il punto nodale è che le risorse debbono provenire da un contenimento della spesa corrente e non da un aumento della pressione fiscale e delle imposte. Ebbene, non è solo una scelta di campo, una scelta di impostazione nei rapporti tra Stato e cittadino, occorre anche misurare le conseguenze sull'economia di un diverso approccio della manovra di politica economica: un conto è aumentare le tasse, un conto è tagliare la spesa. Come con grande onestà intellettuale lo stesso Presidente della Commissione bilancio ha chiarito in Commissione, quando si aumentano le tasse si riduce la crescita economica. Quindi, il primo falso in comunicazione sociale che il Governo sta compiendo nei confronti di tutti i cittadini l'attuale manovra non realizza né il risanamento finanziario, né il sostegno alla crescita economica, né l'operazione di equità fiscale e sociale. Sfido chiunque in quest'Aula a rispondere alle conseguenze che l'applicazione della finanziaria e di questo decreto recheranno sull'economia italiana del prossimo anno. Il Governo ha più volte ribadito uno *slogan* martellante: realizzare questa manovra per avere risanamento, equità e sviluppo. Ebbene, questa manovra, a detta dello stesso Ministro dell'economia, solo per 15 miliardi (dei quali una parte contenuta come prelievo fiscale in questo decreto)

è perché una manovra di 15 miliardi diventa, a detta del Ministro dell'economia, una manovra di 35 miliardi. Larisposta è molto semplice. Si sta attuando un'operazione di spostamento di potere politico sul fronte dell'economia e dei rapporti civili tra Stato e cittadino concentrandolo nelle mani del Governo centrale e in questa operazione si tagliano risorse ai governi locali, all'università e alla ricerca. Questa è l'operazione delineata nei numeri che lo stesso Ministro dell'economia ha ribadito non più tardi dell'altro ieri. Quindi, non stiamo parlando né di un decreto fiscale né di una legge finanziaria, ma di un'operazione che sposta il confine del potere economico e dei rapporti civili tra Stato e cittadino. Si prendono 30 miliardi di euro - 29,5 per l'esattezza - di maggiori entrate fiscali le si collocano dentro i portafogli dei Ministeri del Governo centrale, laddove la volontà discrezionale dei Ministri deciderà come distribuire queste risorse.

anni precedenti è aumentato di 12 punti il peso dello Stato in economia, ma a volte di mezzo punto all'anno. Solo questo anno, rispetto al 2007, aumenta di colpo il confine

legittima sul piano politico, tant'è che in Commissione i colleghi di Rifondazione Comunista hanno rivendicato politicamente questa maggiore intermediazione dello Stato in economia - diventa falsa falsa comunicazione sociale quando non si dice - e sfido a dimostrare il contrario in quest'Aula e fuori - che quest'operazione di aumento della pressione fiscale determina sull'economia italiana le seguenti conseguenze: la ripresa in atto, che darà quest'anno un tasso di crescita pari all'1,7 per cento, verrà uccisa nel 2007 e la crescita economica, a causa di questa manovra, scenderà sotto l'1 Di conseguenza, a causa della frenata che determina questa manovra sull'economa italiana (altro che sostegno allo sviluppo!), si determina

con una previsione di crescita che non incorpora al proprio interno gli effetti negativi e deleteri di questa domanda. Infine, sul piano dell'equità fiscale, se si fanno bene i conti - mi rivolgo ai colleghi della maggioranza - e se non vogliamo prendere in giro la povera gente in questo Paese, sapete meglio di me, facendo bene i conti, che s'introduce un meccanismo fiscale più regressivo dell'attuale e non più progressivo. La piccola iniezione di progressività che si ha attraverso la manovra dell'IRPEF per una fascia di reddito compresa soltanto tra 1.000 e 1.500 euro netti al mese e 1.500 euro netti al mese è fortemente controbilanciata dall'aumento di altri tipi di imposte che sono palesemente regressivi, cioè fanno pagare di più la povera gente. Faccio due esempi: le addizionali locali che, in quanto addizionali, sono regressive. Pagano proporzionalmente di più le fasce di reddito medio e medio - basso. aumento dell'ICI, essendo tale imposta rapportata al valore dell'immobile, evidentemente, a parità di immobile, paga enormemente di più colui che ha un reddito medio-basso. Quindi, da questa vostra manovra esce un sistema fiscale più regressivo e non più progressivo. Questo è l'aspetto economico. Chiudo, Presidente, con l'aspetto dei rapporti civili, come hanno già accennato altri colleghi, perché lo spostamento del confine tra Stato e cittadini non avviene solo in termini di risorse economiche, ma anche in termini di libertà civili. Ha fatto bene il Presidente del Consiglio a lamentarsi di qualcuno che è entrato a mettere il naso nell'anagrafe tributaria e nelle sue dichiarazioni... *(Il microfono

sono trasmesse all'anagrafe tributaria senza alcun criterio di selezione dell'accertamento e senza che si sappia chi abbia titolo

un *vulnus* istituzionale, che ha conseguenze indipendentemente dalla circostanza che nel futuro ci sia al Governo il centro-sinistra o il centro-destra. Abbiamo messo nelle mani di chiunque di chiunque possa accedere con una *password*, falsa o vera, l'intero movimento finanziario e bancario di tutti gli italiani. Con questo decreto applichiamo un altro principio stravolgente, che è quello della retroattività fiscale: in parecchi aspetti di questo decreto si introduce infatti la retroattività delle imposte. Quindi, cari colleghi dell'opposizione, ma soprattutto della maggioranza, riflettete bene sul *vulnus* che stiamo introducendo nella legislazione nazionale di queste materie, perché chiunque sa che il fisco ha sempre avuto la possibilità di accedere ai conti correnti bancari di chiunque, ma ad una condizione: aprire un accertamento e avvertire il contribuente che è sotto accertamento. Si garantisce a tutti un avviso di garanzia, perché non lo si deve garantire a qualunque cittadino italiano che può avere i propri dati a disposizione di chiunque, senza che neanche lui sappia chi va a mettere il naso dentro l'anagrafe tributaria? Nella scorsa legislatura, per un anno e mezzo, abbiamo avuto l'anagrafe tributaria privata

e nella scorsa legislatura abbiamo dovuto ricomprare la società e riportarla nell'ambito del settore pubblico. Questo è ciò che sta avvenendo: false comunicazioni sociali, aumento del peso dello Stato nell'economia, riduzione delle libertà civili di tutti i cittadini italiani (che siano di centro-destra, che siano di centro-sinistra, o che, purtroppo, come vediamo, siano sempre più disinteressati al ruolo centrale e al dominio della politica), con il rischio di lasciare le decisioni ai grandi apparati

la soppressione di commi che introducono quella che, a nostro avviso, è una caratteristica specifica di questa parte del decreto, cioè una sua induzione alla odiosità gratuita, da parte dei cittadini, nei confronti delle istituzioni. Dico ciò perché la caratteristica di questo provvedimento sembra essere quella

il male contrario al presunto bene voluto. Il bene voluto dal provvedimento dovrebbe essere quello di una maggiore contribuzione da parte del cittadino rispetto alla necessità di reperimento di risorse per il miglioramento dell'amministrazione e della finanza pubblica. Ciò che invece si realizza è un'odiosità gratuita, ossia si introducono elementi per cui la doverosità della contribuzione viene garantita attraverso una persecuzione del contribuente. Quali sono gli elementi sostanziali? Essi sono tanti, ma su uno

un cittadino (per un mero refuso o un errore materiale o una pretesa da accertare) abbia nei confronti dello Stato un debito per una cifra superiore a 10.000 euro. Cosa significa questo?

un contribuente è stata emessa una cartella esattoriale per una tassa non pagata, quindi non per un'imposta, per una cifra superiore a 10.000 euro, questi non può ricevere un pagamento. Se, ad esempio, ho

ritorno dell'IVA pagata su di essi (che non ho potuto compensare perché ancora non ho fatturato), di fronte a un accertamento relativo a una tassa da pagare per una cifra superiore a 10.000 euro, dovrò

un significato antievasione, non è possibile che per l'elusione si provveda in un modo assolutamente coercitivo, vessatorio e limitativo della libertà personale, perché non viene ad essere soddisfatta una delle necessità che è la giusta proporzionalità fra il tributo introdotto e il benefico che si ha attraverso quel tributo per la conduzione dell'amministrazione dello Stato. Qual è il motivo per cui si intende limitare assolutamente la libertà del cittadino per perseguire tale finalità? La improporzionalità, il mancato soddisfacimento della proporzionalità a questo punto fa venir meno sia la necessità che la giustezza della finalità.

perché, attraverso il potenziamento della riscossione e delle prerogative degli ufficiali di riscossione, si ha l'introduzione di un sistema giuridico relativo agli accertatori, che non è quello di polizia giudiziaria, e si estendono ad essi certe prerogative con un sistema di persecuzione ancora una volta oltremodo violento e intromissivo negli spazi di libertà del cittadino. Inoltre, a proposito cosa fa il complesso dei commi a cui ci riferiamo e che vogliamo sopprimere? Pensate che, per quanto riguarda la riscossione coattiva - cosa ben differente, come sappiamo, dalla riscossione spontanea

tutte le amministrazioni, per poter realizzare un pagamento inferiore, finiranno per affidare non solo la riscossione coattiva, ma anche la riscossione spontanea. questo se non una limitazione della libera circolazione dei capitali e quindi della concorrenza? Cosa risulta evidente dal complesso di questi commi? Che mentre il Governo, da un lato con il provvedimento Bersani parla di liberalizzazione, dall'altro, con Rutelli, parla di nuove liberalizzazioni dei servizi; dall'altro ancora, con il ministro Mastella (che ringraziamo di essere in Aula, seduto sulla sedia del Presidente del Consiglio a leggere il giornale, onorandoci della sua presenza), si diletta un giorno sì e un giorno no a parlare della liberalizzazione delle professioni;

in esse l'attività invasiva e pervasiva del Governo si è fatta sempre più evidente, con nomine che hanno portato al limite ultimo il concetto e la normativa sullo *spoils system*, se è vero che in questo provvedimento è anche introdotto un sistema per cui non solo si ha la prerogativa da parte del Governo

aumento del gettito fiscale che sta facendo sì che la nuova finanziaria sia costruita non solo sulle vostre scelte, ma sul rinnovato gettito fiscale e sul risparmio, tutti da attribuire al buon governo del passato. Siamo contro queste norme che introducono odiosità gratuita, siamo contro questo provvedimento. È questo il motivo per cui, riservandoci nelle dichiarazioni di voto di continuare ad esporre le motivazioni che ci hanno portato alla presentazione degli sollecitiamo per ora su di essi l'attenzione da parte dei colleghi dell'opposizione.

per due ordini di ragioni: innanzitutto perché, com'è noto, su quel patrimonio sono state preventivamente pagate le imposte sul reddito.

costruito dopo il pagamento delle imposte sui redditi e dunque ritassarlo, a nostro avviso, non è corretto. Ma vi è di più, ne facciamo una questione anche più particolare. Innanzi tutto, in questa norma c'è uno dei difetti cardine di questo decreto-legge, sbagliato nella sua

nel testo del decreto-legge, la questione delle successioni relative ai fratelli; sono presi in considerazione solo i discendenti in linea retta. Tant'è vero che la maggioranza, devo dire un po' simpaticamente, si è esercitata in ordini del giorno che contraddicono il decreto-legge. In particolare, in uno degli ordini del giorno

che si preoccupa di un aspetto particolare, quello della successione nell'impresa di parenti

«Che bell'emendamento ha presentato l'opposizione, è proprio vero, tant'è che faremo un ordine del giorno per sollecitare il Governo a rimediare con una prossima legge». Chiedo scusa, Presidente, se uso qualche parola che può sembrare un po' forte, ma siamo nell'esilarante. Abbiamo qui una norma e la possiamo correggere; no: che forse la correggeremo con una normativa successiva. Non sembri pretestuosa questa mia osservazione. Sotto diversi profili altri colleghi hanno richiamato lo Statuto dei diritti del contribuente, io vorrei richiamarlo sotto un ulteriore profilo. Lo Statuto dei diritti del contribuente imponeva

fare questa correzione». Cosicché il cittadino avrà una norma abrogata in parte e poi modificata e corretta, con un problema di successione delle leggi nel tempo che sarà anche oggetto di contenzioso. Così si fanno norme contorte,

In questo modo state abrogando una legge importante come lo Statuto dei diritti del contribuente e lo fate proponendovi di non farlo. È francamente un modo di fare che sento di dover contestare.

siccome si riferiscono alla variazione della normazione sulle conseguenze della violazione dell'emissione del cosiddetto scontrino fiscale,

sono condivisibili, in quanto fanno parte organica di un ordine del giorno che è stato votato nelle Commissioni che si riferisce allo statuto del contribuente. Evidentemente il parere è contrario per il quarto quarto comma e per la parte di copertura. Quindi è importante il richiamo alle norme dello statuto del contribuente che la maggioranza ha inserito in un ordine del giorno già accolto nei lavori della Commissione.

sull'emendamento 1.27 il parere è negativo perché soppressivo di parti rilevanti dell'articolo 1 del decreto. l'emendamento 1.28, per la parte propositiva che si riferisce alla trasmissione di azienda e quindi alla disciplina delle successioni,

del Governo è conforme a quello espresso dal relatore...

Credo sia utile, signor Presidente, che il parere venga espresso e motivato, per la parte fiscale, dal presidente Benvenuto, per la seconda parte dal sottoscritto.

sta nel fatto che questo decreto, come ammesso anche dalla relazione tecnica, prevede maggiori introiti per la lotta all'elusione e all'evasione fiscale per 4 miliardi di euro, in realtà, non fa una vera lotta all'evasione fiscale, in quanto, solo genericamente e con norme sull'IVA e di controllo, previste nei vari commi di questo articolo, è previsto un vero aggravio fiscale nei confronti del contribuente. Gli studi pubblicati, anche recentemente, da parte di importanti associazioni hanno dimostrato invece come e in quale maniera si svolge il gravissimo fenomeno dell'evasione fiscale in Italia. La distribuzione settoriale e territoriale

a proposito di questo decreto di lotta all'evasione non produrrà nessun tipo di effetto nel senso auspicato. Se, fra un anno o due, andremo

in termini di valore relativo, e i valori assoluti non saranno assolutamente cambiati. Invece troveremo senz'altro cambiato, perché non c'è una politica vera e propria di lotta all'evasione fiscale, e aumentato il carico fiscale nei

che non produrrà altro che un inasprimento fiscale per chi già paga le imposte e che non sortirà alcun effetto concreto e, soprattutto, fattivo - e meno che mai

L'articolo 100, comma 9, del Regolamento recita: «Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati». È chiaro che, all'interno del pronunciamento, c'è la dichiarazione di favore o di contrarietà.

Di qua c'è il partito della libertà, il partito che ha permesso, per dichiarazione nello stesso DPEF

29,4 miliardi in più di entrate, così come è scritto nel bollettino di novembre della Banca d'Italia. Sono dati ufficiali

Perciò intendiamo, proprio con questo emendamento strategico, dire agli italiani e al Paese che c'è una diversa filosofia per risanare i conti dello Stato: di là chi prende, di qua chi libera risorse e consente al cittadino di non avere uno Stato patrigno, ma uno Stato amico. Ecco perché i contribuenti sono emersi naturalmente, volontariamente - sì, cari amici - con i condoni, quei condoni che hanno portato maggiori entrate, senza avere la Guardia di finanza dietro la porta e un commercialista per ogni contribuente. È stata quell'emersione che forse voi non riuscirete mai a ottenere per le ragioni che ho spiegato in discussione generale.

Presidente, voglio dichiarare il nostro convinto voto favorevole all'emendamento 1.3 che - come

già dal 1970, che individua nei diritti del contribuente il presupposto per una sua leale collaborazione con l'amministrazione finanziaria. Questa disposizione prevede una regola basica per l'acquisizione di informazioni relative al contribuente; richiamo l'importanza di questo emendamento anche in relazione alle patologie che sono state recentemente riscontrate negli accessi al sistema dell'amministrazione finanziaria. Proprio ieri il vice ministro Visco ha addirittura proposto una sorta di particolare modalità di accesso alle informazioni contenute nel sistema dell'amministrazione finanziaria per quanto riguarda i contribuenti che egli ritiene più sensibili. I giornali parlano di contribuenti *vip*. Non so come possa definirsi una categoria di questo tipo, cioè una categoria di contribuenti per i quali la tutela dovrebbe essere rafforzata, sembra, nel presupposto che in realtà per i più, per i non *vip*, non esisterebbe un'adeguata tutela relativa alla riservatezza dei dati sensibili che li riguardano. Gli eventi patologici che hanno riguardato numerose personalità hanno, infatti, dimostrato la facilità con la quale non soltanto dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma anche dipendenti della Riscossione S.p.a., e quindi dipendenti del settore privato, possono accedere a questi dati sensibili. Quanto è importante, quindi, riconoscere questo principio fondamentale e uniformare ad esso tutte le disposizioni che lo negano e che sono contenute innanzi tutto in questo provvedimento ma - lo ripeto - anche nel famigerato decreto Bersani-Visco. Sono disposizioni, tutto al contrario, ispirate alla possibilità per l'amministrazione di operare nella assoluta ignoranza da parte del contribuente che si stanno acquisendo valutazioni, oltre che informazioni oggettive, che lo riguardano; valutazioni che egli non avrà mai modo di conoscere e rispetto alle quali non avrà mai modo di opporre le proprie motivate ragioni, che portano a testimoniare la legittimità dei suoi comportamenti. Per questo è importante e basico l'emendamento 1.3, che attiene ad una norma di civiltà. Probabilmente, in quanto tale, una norma di civiltà non sarà votata da questa maggioranza*.

vista l'importanza dell'emendamento 1.3, così come ha spiegato il senatore Sacconi, affinché rimanga agli atti parlamentari la responsabilità di questo voto, chiedo ai colleghi l'appoggio per la votazione

violazioni solo dello Statuto del contribuente, ma, in questo caso, anche della legge sulla *privacy*.È naturale, a questo punto, che il cittadino si trovi completamente con le spalle al muro, sia solo il profilo della temporalità sia sotto il profilo della possibilità di ricevere informazione dell'attività dell'agenzia di riscossione. Quindi non possiamo che chiedere, con l'approvazione dell'emendamento 1.14, soppressivo dei commi 8 e 8-*bis*, che venga corretta questa grave

Signor Presidente, lei ha sostenuto che vi sono diritti e doveri. C'è anche il diritto di chiedere il voto dei senatori a vita oppure no? È stato abolito? PRESIDENTE. I senatori a vita hanno il diritto di votare.

In questo momento stiamo parlando di un emendamento che prevede che si considera evasore fiscale non colui il quale non emette lo scontrino ogni cinque anni, ma colui il quale non lo emette tre volte in un mese. mese. Questa è lotta all'evasione fiscale. Non cade il Governo, anzi probabilmente Visco sarà ancora più contento se passerà un emendamento del genere, perché così si fa seriamente. Vorrei sapere se anche su un emendamento così semplice c'è l'ottusità nel dire di no.

con l'opposizione. La garanzia che i senatori possano votare tranquillamente e liberamente deve essere assicurata dal Presidente

Signor Presidente, vorrei ricordare a molti colleghi, con i quali ho avuto l'onore di collaborare durante la XIII legislatura, che in quella occasione, in cui noi eravamo sempre all'opposizione, varammo un provvedimento di grande levatura

nonostante quella legge preveda talune modalità particolari per la violazione dello Statuto del contribuente, voi insistete a violarlo. Uno dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento in materia tributaria - e la parte tributaria non è certamente secondaria - è proprio

più grave - una valenza retroattiva, mettete in difficoltà proprio i più deboli, coloro che hanno realizzato la loro programmazione economica anche sotto il profilo tributario. Approvare questo emendamento è un atto non solo di civiltà, ma anche di correttezza nei confronti dei 50 milioni di cittadini che ci stanno guardando e che subiranno le conseguenze dell'approvazione di questa norma.

in questo inizio di legislatura il ricorso alle deroghe allo Statuto del contribuente è stato massiccio, tanto che anche i relatori di questo provvedimento ne hanno stigmatizzato

Fa il paio, colleghi senatori, con altri articoli che sono all'interno di questo decreto fiscale che non vanno che nella direzione di fare

ti impedisco la deduzione dei costi degli automezzi, in modo che poi si possa fare un pari e patta fiscalmente ». Quindi, cittadino contribuente, sappi che, se anche ne hai diritto, allo Stato e all'erario non importa niente dei tuoi diritti,

il mantenimento e anzi l'accrescimento dell'evasione totale, perché con la retroattività si va a colpire - come dicevo poco fa - particolarmente, anzi direi esclusivamente chi già è iscritto, chi è già a ruolo e ben conosciuto dall'amministrazione finanziaria.

un inconveniente tecnico. Visto che l'opposizione ha presentato pochi emendamenti sperando in una discussione, non vorremmo che sia stato tolto l'audio al centro-sinistra, poiché nessuno di loro interviene per discutere nel merito dei nostri emendamenti.

dovuto da amministrazioni pubbliche o da società a partecipazione pubblica, per importi superiori a 10.000 euro, qualora il beneficiario risulti destinatario di iscrizione al ruolo. L'esperienza di questi anni non non ci può lasciare tranquilli perché spesso le iscrizioni al ruolo sono risultate erronee o prive di alcuna fondatezza alcuna fondatezza e, tra l'altro, possono essere spesso dovute anche ad un mero refuso, ad un errore materiale o ad una pretesa ancora tutta da accertare.

(come quelle che sono erogate a titolo di trattamento di fine rapporto), con evidenti esiti di arbitraria ingiustizia, che sarebbe così introdotta nel rapporto tributario. tributario. Vorrei ricordare altre disposizioni che vengono abrogate e che riguardano la proposta di compensazione per il contribuente che vanti un rimborso di imposta e, parallelamente, un'iscrizione al ruolo. caso, il meccanismo vale solo ad introdurre odiosi termini dilatori e fasi del tutto artificiose per differire oltre ogni limite di tollerabilità il soddisfacimento di diritti che già sono stati riconosciuti in via definitiva per il contribuente, a fronte di un'iscrizione al ruolo che potrebbe risultare infondata per le ragioni che poco fa ricordavo. Con queste motivazioni - di assoluta tutela del contribuente nei confronti di un comportamento, ancora una volta odioso e quindi discrezionale, da parte dell'amministrazione - il nostro voto, convintamente, è favorevole.

o maggiorazioni di tasse o di imposte che alla chetichella vengono disposte in questo decreto-legge. Per esempio, il comma 45 dell'articolo 2 (del quale chiediamo la soppressione) è quello che rivaluta le rendite catastali nella

l'introduzione, anche in questo campo, di nuove tasse che naturalmente - e direi quasi per inerzia - saranno soggette ad un'estensione della platea dei soggetti che

Una parte degli immobili dei quali viene rivalutata la rendita catastale è quella venduta attraverso le cartolarizzazioni.

saremmo di fronte a fatti certamente di natura civile e probabilmente di natura penale. Noi qui invece lo facciamo alla chetichella, in sordina,

significativo di tali aumenti è che, di per sé, sembrano molto esigui. Si tratta però di 416 euro per 1.000 litri di prodotto

qualche piccola aliquota di IRPEF, ricordate bene a quegli stessi cittadini che già da ora abbiamo aumentato il gasolio. Il gasolio

che abbiano quasi un carattere di vessatorietà, perché è evidente che che penalizzare coloro che usano l'autoveicolo o comunque il mezzo a trazione con combustibile per lavoro significa contribuire ad uno dei pericoli che ho paventato in altri interventi, ossia contrastare sul nascere il processo di crescita economica che ha accompagnato l'Italia in questi mesi. Chiedo pertanto che tali norme vengano riviste e che si voti favorevolmente all'accoglimento dell'emendamento

il tema ampiamente trattato, sia in campagna elettorale sia negli ultimi tempi per la predisposizione della legge finanziaria e del decreto collegato, dell'imposta di successione.

«La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che nell'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di successioni e donazioni si escludano le situazioni in cui il beneficiario

per la cessione di quei rami d'azienda, in specie nel settore agricolo, dove l'impresa, cioè la personalità giuridica, è coincidente con la persona fisica.

è naturalmente a favore dell'emendamento 1.28, che rappresenta una questione centrale sulla quale abbiamo chiesto una modifica. La maggioranza non si può rifugiare, come ha fatto, negli ordini del giorno. Ho contato 178 impegni di modifica. Questa è la dimostrazione che occorre intervenire con correzione profonde. Noi abbiamo posto un problema con questo emendamento,

Abbiamo bisogno di sindacalisti? Forse sì, perché molti fanno carriera. Crediamo però che questo Paese abbia bisogno di imprenditori e di aziende,

Presidente, per questi emendamenti vale ciò che ho detto prima. Molti di essi sono emendamenti presentati dall'intera opposizione, quindi spero di riuscire ad illustrarli tutti.

la stessa configurazione dell'emendamento 1.100 e, per quel che mi riguarda, l'ho già illustrato. In dichiarazione di voto si potrà ritornare sull'argomento al quale diamo, come opposizione, grande importanza perché si tratta di delineare, seppur sommariamente, una manovra alternativa a quella proposta dal Governo. Mi soffermo invece su un emendamento sul quale abbiamo insistito in campagna elettorale, quello che riguarda l'abrogazione dell'ICI sulla prima casa. Molti avevano ritenuto che fosse una trovata elettorale del presidente Berlusconi. Con l'emendamento 2.850 vogliamo mostrare, e crediamo di esserci riusciti, che quella, invece, era una seria proposta di riduzione delle tasse a favore di una fascia di cittadini che noi riteniamo determinante (coloro i quali sono riusciti ad acquistare una prima casa nella loro vita) e che avrebbe potuto costituire un segnale serio di riavvicinamento tra il fisco e i cittadini.

perché le polemiche che furono fatte erano del tutto fuori luogo. Sosteneva il presidente Berlusconi che si trattasse di una grandezza assolutamente padroneggiabile nell'ambito degli strumenti di copertura della legge finanziaria e/o del bilancio. Noi, con questo emendamento, lo dimostriamo. Cosicché quella proposta, che a molti parve mera questione elettorale, per noi è invece proposta praticabile e meritevole di accoglimento.

voglio soltanto ricordare un aspetto che da molti non è stato ancora adeguatamente sviluppato: i poteri abnormi

a questo proposito, il comma 8 dell'articolo 2: «Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Siamo fuori da ogni logica. All'esattore è concesso di violare ciò che talvolta non è concesso di violare nemmeno al giudice. Ora, io auspico che almeno queste norme, che rappresentano un grado di vessatorietà fuori da ogni limite, siano modificate in questa lettura, da questa Camera, con questo provvedimento. Ci soffermeremo su tali questioni, ma mi è parso opportuno, in sede di illustrazione, gettare l'allarme su di esse. Siamo di fronte all'invasività del potere tributario al di là di ogni limite accettabile. Se non poniamo, qui ed ora, un freno a questo atteggiamento dello Stato fiscale nei confronti del cittadino inevitabilmente ci troveremo di fronte ad un contenzioso pesante e a nuove forme di tentativi di evasione. Noi, invece, siamo per riportare alla correttezza il rapporto tra Stato e cittadino, perché solo in questo modo si combatte efficacemente l'evasione. [FRANCO

Prego, senatore

la questione dell'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili da parte del concessionario delle riscossioni, mentre il fermo amministrativo. Abbiamo presentato degli emendamenti con dei commi aggiuntivi perché, all'interno del decreto fiscale, si tratta del problema della riscossione. Come ho già accennato prima,

in termini poveri, è assolutamente disarmato nei confronti di chi procede coattivamente a questa riscossione. Come l'esperienza ci ha insegnato negli ultimi anni a mezzo stampa, a mezzo indagini o a mezzo interrogazioni, interrogazioni, spesso e volentieri ciò accade senza giustificato motivo, con errori che non vanno che nella direzione di rendere assolutamente impotente il cittadino a difendersi nei confronti dei concessionari della riscossione.

Il comma 18 dell'articolo 2 prevede, sostanzialmente, un'eliminazione di questo tipo di ammortamento,

vi è un incremento del costo delle diverse deduzioni a parte delle imprese. Quindi, anche in questo caso abbiamo proposto, con

ricordare l'importanza che ha nel rapporto, questa volta non tra Stato e cittadino, ma tra Stato e enti locali, nel momento in cui andiamo a trattare dell'ICI:

2.41 prevede l'abrogazione dei commi 71 e 72 dell'articolo 2 che tratta delle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati in esercizio di imprese, arti e professioni.

chiede di modificare le percentuali (che sono state ridotte) di deducibilità, secondo quanto è stato previsto nel decreto-legge a modifica del testo unico delle imposte sui redditi, e di renderle meno penalizzanti

rivolta alle società di capitale pubblico e alle amministrazioni pubbliche, di non effettuare versamenti per importi superiori a 10.000 euro, nel caso venga accertato che esiste contenzioso contenzioso o non pagamento di cartelle erariali normalmente notificate al soggetto fiscale, al soggetto d'imposta. Vi è quindi l'obbligo, ove

di non procedere al pagamento del creditore, fornitore di beni o di servizi, e di segnalare all'agente della riscossione la circostanza, al fine di consentire all'agente medesimo di procedere al recupero delle somme. Signor Presidente,

Ci troviamo, in base a questa previsione, di fronte ad una serie di incongruenze. Innanzi tutto, la norma è rivolta ai soggetti d'imposta che siano enti pubblici o società con capitale pubblico. Ma perché non anche alle società private, allora? Soggetto d'imposta l'uno, soggetto d'imposta l'altra. l'altra. Siamo di fronte ad un atteggiamento di discriminazione di trattamento dei due soggetti giuridici d'imposta a seconda che siano pubblici o con capitale pubblico, oppure società di diritto privato. privato. Ma vi è anche un aggravio di responsabilità e di costi per i soggetti pubblici o per le persone giuridiche pubbliche, in quanto si fa loro carico di quell'accertamento preventivo che, viceversa, il soggetto privato non ha. Si introduce, signor Presidente, signor relatore - e noi crediamo proprio che condizioni di ragionevolezza dovrebbero indurvi ad accogliere, ringraziandoci, il suggerimento che vi stiamo dando in senso

che, avendo soltanto opposto una cartella erariale regolarmente notificatagli per oltre 10.000 euro, non ha diritto a veder pagati i propri crediti di fornitura, vuoi dalle Ferrovie dello Stato, vuoi da Alitalia? Alitalia? Porremmo queste società in una condizione di grave e accentuata difficoltà; indurremmo, cioè, i fornitori di beni o di servizi per queste società a riflettere e ripensare mille e una volta

ci appelliamo alla sensibilità e al senso di responsabilità dei colleghi della maggioranza, tener conto di questa segnalazione e di questa nostra richiesta di sopprimere la norma in questione.

in seconda lettura si procede unicamente all'accertamento preliminare della conformità della copertura del disegno di legge finanziaria alle regole stabilite in questa materia dalla vigente legislazione contabile. Ciò premesso, sentito il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato e preso atto anche della posizione assunta in materia dal Governo, comunico le determinazioni della Presidenza che prego il senatore segretario di leggere all'Assemblea. «Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2007 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468 del 2006, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. Si segnala al riguardo che anche nella sessione di bilancio 2007-2009 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti

n. 1183), dal momento che dall'allegato recante lo schema di copertura si desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2007 rientrano, per gli importi recati dal relativo prospetto, anche le maggiori entrate di cui al citato decreto-legge. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2007-2011 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2007) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti leggermente inferiore all'obiettivo fissato nella predetta Nota ed è pari a 29 miliardi. Per il 2008 e 2009 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, in linea quindi con l'indicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2007-2011, ancorché superiori in termini assoluti; poiché però i vincoli per il secondo e terzo anno sono stati posti dalla citata risoluzione come tappe di avvicinamento agli obiettivi programmatici, il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2007-2009, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2007. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute dei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata».

i disegni di legge n. 1183 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e n. 1184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009); conseguentemente le Commissioni sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi.

della seduta inaugurale di questo ramo del Parlamento, pronunciate dalla senatrice Finocchiaro che, facendo riferimento alla necessità di operare in quest'Aula secondo criteri di rigorosa eticità politica, diceva che bisogna rifarsi ai richiami e alle indicazioni di Max Weber. Anch'io, signor Presidente, come avrà dedotto dal testo della lettera che le ho fatto pervenire in via informale e preventiva, uso, nei miei atteggiamenti e nei miei comportamenti, esercitare e muovermi in un rigore sistematico e soprattutto con quell'impegno

le prospettive e i cammini più sicuri, più luminosi e certi. Noi siamo chiamati a realizzare le cose più certe, più sicure e più altamente democratiche. Allora, presidente Marini,

di contare sulla sua sensibilità altamente democratica, da lei corrisposta con la sua replica, breve ma efficace, alla mia lettera. Ebbene, signor Presidente,

tutti i membri di quest'Aula del testo della mia lettera e della sua risposta, in modo da evitare per un verso di tediare i pochi volenterosi presenti - altri

nell'iniziativa - di accademici costituzionalisti, di tecnici della pubblica amministrazione e della contabilità generale dello Stato e del bilancio pubblico,

Tutti sono stati concordi nell'affermare che i rilievi da me mossi e le perplessità da me sottoposte, signor Presidente, hanno totale e assoluta fondatezza. Il *vulnus* di cui parlo è quello relativo all'ex articolo 53 del testo discusso alla Camera, che investe - questo le segnalo nella mia lettera - aspetti di legittimità, di legalità e di costituzionalità. Signor Presidente, anche su sua cortese sollecitazione, questa mattina mi sono recato presso la Commissione bilancio accolto con delicatezza e generosità, mi è stato consentito, finanche in oltre venti minuti, di esporre alla Commissione le ragioni della mia preoccupazione. È stato però agevole per il Presidente della Commissione dire - e anch'io forse avrei fatto altrettanto

opera di salvaguardia delle prerogative di questo ramo del Parlamento. Io non ho il minimo dubbio delle sue alte qualità,

gravità, per quanto - ripeto - mi è stato certificato da specialisti sia del ramo giuridico-costituzionale sia del ramo tecnico-contabile dello Stato, affermo

in una circostanza così traducibile: lei è alla guida del convoglio, del convoglio, che è questa Camera; quest'Assemblea ha le ruote ed un volante. Lei ha tutta la responsabilità tutto il diritto-dovere di guidare il convoglio come ritiene vada guidato, secondo le sue prerogative e le sue facoltà. durante la sua guida qualcuno le segnala che quella direzione

«le mie prerogative sono queste e vado dove voglio, finanche nel fossato». Lei deve interpellare gli specialisti di guida,

di sospendere l'introduzione nell'Aula e nelle Commissioni di questo disegno di legge. La ringrazio; veramente, e le sono grato, signor Presidente, per la possibilità che mi ha

È stato letto il parere, dopodiché dovrebbe seguire la dichiarazione del Presidente per l'apertura della sessione di bilancio, sentito il parere della 5a Commissione. È d'uso, non previsto dal Regolamento, che sulle comunicazioni fatte all'Assemblea per il parere espresso alla 5a Commissione ci sia un intervento da parte di coloro che in Commissione hanno fatto osservazioni e che per il voto di maggioranza non sono state ricevute all'interno del parere. A questo intervento sta preparandosi il senatore Azzollini, ma è chiaro che all'ora alla quale ci troviamo questo intervento del Presidente non ha la possibilità di essere ascoltato non soltanto dal Parlamento, ma anche dai rappresentanti della maggioranza che sono stati maggiormente impegnati nella redazione del provvedimento, e per primo il Presidente della Commissione bilancio. Proporrei

le questioni trattate, che riguardano, come abbiamo più volte detto nel corso dei lavori, un tema rilevante per il dibattito politico rilevante, cioè la trattazione e trasformazione della legge finanziaria e della legge di contabilità.

e non ce ne voglia il Sottosegretario, che ha seguito i lavori in Commissione. La sessione di bilancio è disciplinata molto correttamente. Probabilmente, andremo verso una riforma

la prassi, che vuole che i giudizi di ammissibilità, di legittimità costituzionale, di copertura finanziaria (insomma, tutti gli aspetti definiti dall'altro ramo del Parlamento